hanno avanzato, ai sensi dell’articolo 5, comma 2-bis, del Regolamento, la richiesta di procedere all’elezione di ulteriori senatori Segretari. Il Consiglio di Presidenza, nella riunione del 5 aprile scorso, ha accolto tale richiesta. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2-ter, del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un solo nominativo. Risulteranno eletti i due senatori iscritti ai Gruppi, la cui richiesta è stata accolta dal Consiglio di Presidenza, che otterranno il maggior numero di voti, limitatamente a un senatore per ciascun Gruppo richiedente. Per garantire il più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, davanti al banco della Presidenza è stata approntata una cabina. I colleghi senatori, immediatamente prima dell’ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari una scheda

e obbliga noi tutti all’azione politica affinché l’utilizzo delle armi chimiche contro i civili sia immediatamente fermato. Si devono condannare con forza e compattezza internazionale gli autori e i mandanti di tali scellerate azioni. Non può esistere alcuna attenuante di fronte a tanta cieca violenza, che ci ricorda - ahimè - da vicino le stragi di civili che colpirono il centro Italia per mano dei nazifascisti alla fine della Seconda guerra mondiale. Signor Presidente, ci permettiamo, tramite la Presidenza del Senato, di richiedere con forza e immediatezza la presenza del Governo in quest’Aula per riferire sulle azioni che stiamo perseguendo nelle apposite sedi istituzionali e internazionali. Chiedo che si dia urgenza alla richiesta di presenza del Governo su questa questione di politica internazionale così importante e che ci sta molto a cuore. (Applausi dai Gruppi PD e

Signor Presidente, colleghi, in Siria c’è una guerra si protrae ormai dal 2011. In sette anni sono morte centinaia di migliaia di persone. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, si contano circa 7.600.000 7.600.000 sfollati interni e oltre 5 milioni di rifugiati all’estero. La Siria era un Paese bellissimo; oggi è un Paese che rischia di scomparire. Da tempo è diventato una polveriera. Il territorio è spartito tra milizie jihadiste, lo “stato islamico” e forze ribelli antigovernative, mentre alcune aree sono ancora sotto il controllo del regime di Damasco. Quella in corso è, evidentemente, una guerra per procura, giocata, da una parte, da Mosca e Teheran a sostegno del regime di Assad e, dall’altra, da Stati Uniti e Arabia Saudita, che da tempo puntano a rovesciare il regime. La principale vittima di tutto questo caos, purtroppo, è stato ed è ancora oggi il popolo siriano. Ebbene, in queste ore stiamo registrando un’escalation di tensione che ci preoccupa: prima l’attacco chimico di Douma, una strage terribile, che segue ulteriori attacchi chimici già commessi in passato nel Paese - ricordiamo tutti, purtroppo, Ghuta nel 2013 - e, anche in questo caso, lo scambio di accuse tra le parti in causa è stato immediato. Poche ore più tardi, poi, il botta e risposta a colpi di tweet, con il presidente americano Donald Trump che ha minacciato una risposta dura in Siria, attraverso missili belli, nuovi e intelligenti e la Russia, che si è detta pronta ad abbatterli tutti. I toni, di per sé, come ho già detto, suscitano enormi preoccupazioni. Sembra che lo scenario stia cambiando velocemente e l’ipotesi di un intervento nel Paese appare, purtroppo, sempre più concreta. Alla luce di tutto ciò, in questa fase assai delicata e complessa, riteniamo che il presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni Silveri debba quanto prima informare il Senato sugli sviluppi in corso, soprattutto in virtù dell’esito elettorale del voto del 4 marzo e della nuova composizione parlamentare in essere. (Applausi Signor Presidente, la situazione in Siria non può che suscitare preoccupazione, a cominciare dalla guerra, che è in corso da parecchi anni, ma l’evoluzione che c’è stata in questi ultimi giorni deve metterci in particolare allerta. La questione dell’attacco chimico va approfondita, in ogni caso va fatta chiarezza sull’episodio se c’è stato un attacco chimico, bisogna indubbiamente prenderne atto e adottare delle contromisure. Ma bisogna anche prendere atto dell’escalation che c’è in questi giorni e del pericolo di un conflitto armato esteso a potenze al di fuori del territorio siriano, con conseguenze sugli equilibri e sulla stabilità dell’intero Mediterraneo. L’Italia, per la sua posizione, per la sua storia e per il suo ruolo politico deve avere un ruolo in questa fase, deve far sentire la propria voce e deve lavorare per evitare

Per questo motivo mi associo a quanto hanno detto prima di me i presidenti Marcucci e Toninelli, nel chiedere che il Governo riferisca all’Assemblea e venga in Aula per affrontare la questione, che è estremamente importante, indipendentemente dal momento politico interno, evidentemente,

Signor Presidente, in queste ore i nostri elettori, i cittadini italiani, sono molto preoccupati per lo svolgersi degli avvenimenti in Siria e anche perché hanno una sensazione molto sgradevole, cioè quella di assistere a un film per molti versi già visto: credo che tutti noi ricordiamo l’immagine estremamente iconica, come oggi si suol dire, di Colin Powell con la sua fialetta e quasi tutti noi - forse un po’ di meno - ricordiamo Tony Blair, quando chiese scusa ai suoi elettori per aver sostenuto l’attacco contro l’Iraq, del quale i suoi servizi avevano detto che deteneva nocive e letali armi di distruzione di massa, che poi in effetti non vennero trovate. Quindi mi associo innanzitutto alle parole del senatore Malan, nell’esortare alla prudenza e nel portare avanti l’esigenza di conoscere ed appurare esattamente i fatti prima di deliberare. Il rischio di un’escalation è estremamente serio e mi chiedo, in tutto questo scenario, quale sia il ruolo di quell’Unione europea, più comunemente nel nostro dibattito chiamata impropriamente Europa, che viene da molte parti politiche sostenuta proprio sulla base dell’argomento che sarebbe un interlocutore autorevole che sarebbe capace di intervenire e di gestire situazioni di conflitto geopolitico, come quella alla quale stiamo assistendo. Basta pensare al precedente della Libia: in che cosa ci ha aiutato la nostra fratellanza europea? Abbiamo avuto la sensazione di essere traditi e abbiamo anche avuto, non la sensazione, ma l’evidenza del fatto che sconvolgere equilibri geopolitici da noi non da noi non pienamente compresi ha determinato una catastrofe umanitaria, che poi si è riflettuta in modo molto pesante sulla vita degli italiani con il fenomeno dei flussi migratori, creando tanti rifugiati, tante tante persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Non dobbiamo mai dimenticare che a monte di tale situazione drammatica ci sono state scelte di carattere politico e in particolare militare che poi si sono rivelate avventate. Questo è un rischio che noi non possiamo permetterci di correre, dovendo ancora sopportare le conseguenze di precedenti scelte avventate e per questo mi associo a chi mi ha preceduto nel chiedere che il Governo venga a riferire in Aula, venga ad informarci e soprattutto a dirci di quali informazioni realmente dispone e che cosa sta chiedendo nelle sedi competenti perché venga fatta, con un’inchiesta internazionale indipendente, luce su quanto realmente accaduto. (Applausi

Presidente, in queste ore il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato un probabile attacco missilistico contro la Siria per punire il gravissimo attacco chimico avvenuto nella città di Douma da parte del regime siriano e, secondo le parole presidente Trump, di quell’«animale di Assad». È stata stabilita la pena, non è stata ancora provata la colpa, posto che gli ispettori internazionali dell’ONU non si sono ancora espressi circa il presunto attacco chimico che c’è stato nella città di Douma, sulla natura dell’attacco e sui responsabili dello stesso. Di fronte a una situazione che potrebbe velocemente degenerare, con conseguenze inaspettate per tutta l’area mediorientale e di conseguenza per quello che può accadere in Europa, si consiglierebbe quanto meno il minimo di prudenza necessario a stabilire esattamente cosa è accaduto e chi sono i responsabili.

questo motivo, come Gruppo Fratelli d’Italia, chiediamo che il Governo agisca in ogni sede possibile affinché qualunque atto compiuto a livello internazionale sia valutato con la dovuta attenzione e siano impedite azioni avventate come quelle che sembrerebbero in procinto di essere commesse.

è ovvio che anche noi chiediamo con forza, per dare anche un senso e una compostezza istituzionale alla nostra discussione,

avere contezza delle informazioni e di come il Governo ancora in carica intenda muoversi. Vede, signor Presidente, credo che la cosa più importante in questo momento sia fermare l’escalation, prima che inneschi conflitti dall’esito potenzialmente devastante sia sullo scenario mediorientale, sia su quello più generale, con il rischio, che mi pare molto serio, di un fronteggiamento tra USA e Russia. L’uso di armi chimiche è una cosa gravissima: tutti noi siamo sgomenti davanti alle immagini di quello che è accaduto e che sta accadendo e certamente bisogna, con determinazione e - aggiungo - con certezza, individuare

i più elementari diritti umani e si è fatto anche strame della legalità internazionale. La Siria, purtroppo, è diventata un campo di battaglia nel quale, a spese della popolazione civile (questa è la costante), sono intervenute pesantemente tutte le potenze straniere (Iran, Turchia, Russia, Israele, USA) non per cercare una mediazione capace di salvare migliaia e migliaia di vite di civili, ma solo per appoggiare una fazione contro l’altra. Voglio soltanto qui ricordare i curdi, che sono stati prima esaltati dall’Occidente come eroi della libertà e poi ignobilmente abbandonati e sacrificati sull’altare della Realpolitik. Il mondo ha per anni guardato da un’altra parte, senza rendersi conto che la crisi siriana, senza più alcun controllo internazionale, si stava trasformando in una minaccia per tutti. Devo dire che proprio in questo silenzio assordante colpisce anche l’impotenza totale e l’assenza dell’Unione europea, della non abbiamo quasi nessun cenno, nessun elemento. Eppure sapete perfettamente quanto proprio la crisi e la Siria in un campo di battaglia abbia conseguenze dirette non solo sugli equilibri internazionali, ma anche direttamente sul nostro Paese. cui la situazione sta diventando ancora più deflagrante e rischia di trasformarsi in un conflitto dagli esiti assolutamente

in qualche modo a spingere il Governo a intervenire in senso positivo per quel territorio. Purtroppo, anche noi dobbiamo sottolineare come ancora una volta ci sia il silenzio assordante dell’Unione europea e credo che questo sia uno

Presidente, colleghi, sono un portavoce del popolo campano. Colgo l’occasione per portare all’attenzione di quest’Aula le preoccupazioni di centinaia di lavoratori dei punti vendita Auchan Napoli e, più in generale, di tutti i lavoratori dei punti vendita della Campania. Mugnano, Giugliano, Nola e Pompei stanno vivendo in queste ore momenti di grande preoccupazione circa il proprio futuro. A quanto pare, già a fine mese il famoso marchio francese chiuderebbe i battenti, così come è appena avvenuto a Catania (La Rena). Siamo solidali con gli amici catanesi. 11 Aprile 2018 Non è possibile, Presidente! Lo dico da napoletano, ma soprattutto lo dico da ex-dipendente Auchan. Martedì 3 aprile 2018, alle ore 8 circa, l’azienda Auchan retail Italia, comunicava ai lavoratori del centro commerciale Auchan Napoli (Via Argine) che l’azienda avrebbe interrotto l’attività lavorativa nel corso del mese corrente, creando panico, sconforto e delusione tra i dipendenti. La nota aziendale comunicava inoltre: «Con senso di responsabilità l’azienda è impegnata a limitare gli impatti sociali, cercando di individuare le migliori soluzioni per ogni collaboratore». Peccato che della nota si evinca che questa operazione potrà garantire continuità occupazionale solo per una parte dell’organico; si deduce, quindi, che il posto di lavoro non sarebbe assicurato a tutti e che alcuni rimarrebbero senza. Altri lavoratori ancora ci dicevano che le condizioni contrattuali non sarebbero state le stesse. Sempre nella nota stampa si legge: «Nonostante gli sforzi dell’azienda per il rilancio commerciale dei due punti vendita, la situazione di questi due ipermercati non è più sostenibile». Ma ci si dimentica di dire che, nonostante gli sforzi dei dipendenti, che con senso di responsabilità hanno sempre dato tanto all’azienda adattandosi alle numerose numerose esigenze che gli si chiedevano, questi sono stati trattati come persone sconosciute. E gli sforzi che lo Stato ha fatto per l’azienda? Con il collega del Movimento 5 Stelle alla Camera, Andrea Caso, ci siamo recati personalmente in questi punti vendita; abbiamo parlato con i lavoratori e raccolto le loro sofferenze: pianti di commozione di padri e madri con figli a carico disoccupati o studenti da mantenere. A mio avviso, questa non è una cessione di ramo d’azienda, Presidente: questa è una speculazione commerciale! Signor Presidente, invito a prendere a cuore le sorti di questi lavoratori; sarebbe il caso di convocare i vertici per ricevere le opportune rassicurazioni, soprattutto per avere spiegazioni circa l’utilizzo dei fondi statali e quale piano industriale sia stato applicato oltre al progetto denominato «Discount Italia Sud». (Applausi